del 26 luglio 2012,

Onorevoli colleghi, come purtroppo è tristemente noto a tutti voi, anche stamane in Francia persone innocenti sono rimaste vittima della violenza terroristica. L'episodio questa volta è accaduto in una chiesa vicino Rouen durante la messa del mattino. Le autorità competenti stanno ancora compiendo i necessari accertamenti. Lascia sgomenti il fatto che, nel cuore dell'Europa,

è stata teatro di attacchi e violenze, che ci hanno scosso nel profondo: prima un'aggressione a colpi d'ascia su un treno regionale, poi la strage degli adolescenti nel centro commerciale di Monaco, quindi l'attentato suicida di Ansbach in occasione di un concerto. Si tratta di fatti che si susseguono senza tregua e l'Europa, ma anche altri Paesi extraeuropei, sembrano colpiti da un vortice di aggressione violenta, quasi a voler scardinare i fondamenti di civiltà e di pace sui quali poggia la nostra storia e su cui vogliamo che si fondi anche il nostro futuro. A Kabul, tre giorni fa, un attentato terroristico ha causato almeno 80 morti e oltre 230 feriti, mentre vanno oltre ogni immaginabile orrore le notizie che provengono dagli scenari di guerra e che questa volta riguardano fatti veramente inaccettabili, come i bombardamenti miranti esplicitamente a colpire ospedali pediatrici. L'ingiustificabile violenza che ha colpito i luoghi di aggregazione e di preghiera investe tutti noi, sconvolge i nostri sentimenti e disorienta tutti i cittadini europei. In questi giorni di dolore e di sgomento, il Senato è vicino alle istituzioni e ai cittadini di tutti i Paesi colpiti. Nell'esprimere il cordoglio della nostra Assemblea per tutte le vittime di questa feroce violenza, invito ad osservare un minuto di silenzio.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, la relazione del provvedimento in esame, per la parte di mia competenza, riferisce degli aspetti legati alle obbligazioni finanziarie e contrattuali, a partire dall'articolo 1, comma 1, dove si interviene relativamente alla restituzione del prestito di 300 milioni di euro da parte dell'amministrazione straordinaria. Al riguardo, si ricorda che il decreto-legge n. 191 del 2015 aveva disposto l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, «indispensabile per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria», ossia per permettere alla gestione straordinaria di continuare l'attività produttiva, ovvero per consentire di provvedere al pagamento degli stipendi, dei fornitori e della manutenzione. All'indomani dell'adozione del decreto-legge n. 191, la Commissione europea avviò un'indagine approfondita per stabilire se il sostegno dello Stato italiano alle acciaierie ILVA rispettasse o meno la normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato: un'indagine estesa anche al prestito di 300 milioni di euro. Tale normativa, infatti, non consente l'erogazione di sostegno pubblico per correre in soccorso e avviare una ristrutturazione delle imprese che versano in difficoltà. La siderurgia è stata esclusa da questo tipo di aiuti a metà degli anni Novanta, di comune accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione.

consente agli Stati membri di erogare aiuti volti a migliorare la competitività delle acciaierie europee su scala mondiale, ad esempio, ai fini di ricerca e sviluppo, formazione e sostegno alle attività ad alta intensità energetica. Così negli ultimi anni i vari Stati membri hanno adottato misure tese a compensare, per gli elevati costi che si trovano a sostenere, quelle industrie che svolgono attività ad alta intensità energetica, tra cui le acciaierie. Sebbene influiscano sulla concorrenza nel settore siderurgico, infatti, queste misure promuovono importanti obiettivi di interesse comune. Il Governo italiano ha chiesto più volte di rivedere l'intero regime degli aiuti di Stato per il settore dell'acciaio. La modifica che intercorre nel decreto-legge in esame va proprio a intervenire relativamente a quanto ci è stato chiesto dalla Commissione europea. Nel testo precedente, infatti, si disponeva che fosse l'aggiudicatario della procedura a provvedere alla restituzione allo Stato dell'importo di 300 milioni maggiorato con gli interessi; con le modifiche introdotte, invece, l'obbligo di restituzione dei 300 milioni erogati dallo Stato è posto a carico dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA, a cui tali somme sono state effettivamente corrisposte, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cessazione dell'impresa, anteponendolo ad altri crediti. Tale modifica assicura la discontinuità, anche economica, della gestione da parte dei soggetti aggiudicatari ed è in linea con le indicazioni della Commissione europea, che, anche con la *comfort letter* relativa alla procedura di vendita in corso, ha ribadito che la restituzione in capo all'aggiudicatario pregiudicherebbe il conseguimento della discontinuità economica tra cedente e cessionario. Sulle modifiche alla procedura di aggiudicazione un aspetto importante, che sottolineo, è che tali modifiche legano strettamente il piano industriale a quello ambientale. Tra i vari aspetti, frutto del dibattito avvenuto alla Camera, vi è l'obbligatorietà per gli aggiudicatari di inviare ogni sei mesi una relazione sull'attività posta in essere riguardo al piano ambientale e rispetto alle obbligazioni contrattuali. Questo al fine di garantire una maggiore trasparenza da parte dell'aggiudicatario nella gestione sia del piano di risanamento ambientale, sia del piano industriale. Sempre al comma 1 dell'articolo 1, va sottolineata una modifica alla disposizione che disciplina la procedibilità dei crediti, allo scopo di dare priorità al pagamento dei debiti ILVA nei confronti delle piccole e medie imprese dell'indotto.

nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario. Va inoltre sottolineata la modifica che stabilisce che le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario, dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Il comma 2 dell'articolo 1 interviene in materia di affitto di azienda o di rami di questa, con obbligo di acquisto nell'ambito della procedura di cessione dei complessi aziendali. In particolare, si prevede che la disciplina dettata dalla legge fallimentare non si applichi qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'affittuario; dunque non è prevista l'ispezione dell'azienda, né il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria, né il diritto di prelazione dell'affittuario. Resta fermo, in base alla norma, l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni del medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge. Per dare certezza alla prosecuzione dell'attività produttiva per affittuari o acquirenti, l'articolo 1, comma 3, novella l'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», al fine di estendere all'affittuario o all'acquirente dei complessi aziendali ILVA l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e la conseguente commercializzazione dei prodotti. Si ricorda in proposito che l'innovazione introdotta dal decreto-legge n. 207 del 2012 è stata quella di consentire, a seguito dei provvedimenti di sequestro disposti nei confronti di ILVA dall'autorità giudiziaria, la prosecuzione dell'attività produttiva per un tempo determinato in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, vincolandola a taluni presupposti: l'accertamento dell'assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione, essendo l'attività esercitata in uno stabilimento di interesse strategico-nazionale, nonché la tutela dell'ambiente e della salute. reca disposizioni in merito ai finanziamenti ad imprese strategiche. In particolare, il comma 1 dispone che gli importi dei finanziamenti statali concessi ai commissari del Gruppo ILVA siano rimborsati non più nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati (800 milioni, di cui 600 nel 2016 e 200 nel 2017), bensì nell'anno 2018, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, stabilita nella medesima disposizione. Il comma 2 dell'articolo 2 provvede agli oneri di cui al precedente comma, in termini di fabbisogno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a compensazione del quale si prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali, su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero (la cassa per i servizi energetici ambientali è un ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua). Il comma 3, sempre dell'articolo 2, stabilisce che agli oneri derivanti dai maggiori interessi passivi, di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. signora Presidente, onorevoli colleghi, continuo a pensare quanto sia demagogica e strumentale la posizione di chi si distingue sulla linea di non intervenire sul complesso aziendale ILVA. La retorica dei dieci o degli undici decreti non appartiene ad una forza di Governo che antepone questioni ambientali e di rilancio di un così importante complesso industriale, oltre che dell'impatto sull'occupazione e sulle piccole e medie imprese coinvolte, in un territorio che invece ha bisogno della determinazione risolutiva, consci che l'industria siderurgica possa e debba svolgere un ruolo fondamentale, praticata nel rispetto dell'ambiente e della salute, per lo sviluppo economico complessivo

le Commissioni riunite 10a e 13a propongono oggi all'Assemblea la conversione in legge di un decreto-legge sull'ILVA che, a nostro avviso, risulta notevolmente migliorato rispetto al testo originario presentato dal Governo. Il ricorso a un ulteriore decreto-legge è a questo punto inevitabile per garantire il proseguo dell'attività economica di un importante stabilimento a livello nazionale e, al contempo, provvedere a un risanamento ambientale serio e realisticamente possibile, che le procedure esistenti non avrebbero potuto consentire. Difatti, troppo complesse erano e rimangono le problematiche lasciate in eredità dal gruppo Riva. Da questa considerazione si sono sviluppate le numerose deroghe alle norme ordinarie in campo ambientale e giuridico che troviamo in diversi di questi decreti-legge; tutto questo in una situazione - lo ricordo - di crisi economica che ha investito la siderurgia mondiale, in una situazione di competitività molto accesa. Difficilmente si sarebbe potuta intraprendere un'altra strada. Si sarebbe potuto chiudere, o meglio far chiudere, gli stabilimenti ILVA, una scelta che, a nostro avviso, è assolutamente da evitare, non solo per una questione occupazionale, sicuramente molto importante, ma per le gravi implicazioni ambientali che tale decisione comporterebbe. Il nostro Paese è, purtroppo, pieno di situazioni che hanno prodotto siti cosiddetti «orfani»: si pensi, solo per citarne uno, alla vicenda della Caffaro, che ha riguardato Torviscosa, la Valle del Sacco, Brescia, che ci ha lasciato in eredità centinaia di ettari e vaste aree di falde contaminate, che richiedono centinaia di milioni di euro per essere bonificate, che ricadono inevitabilmente sulle spalle del pubblico e che continuano a costituire un serio pericolo ambientale. Un percorso, quindi, quello scelto, coraggioso, sicuramente sofferto, che presenta delle situazioni discutibili, ma a nostro giudizio, in questa fase, assolutamente inevitabile. Ricordo, preliminarmente, che il decreto-legge al nostro esame, che consta ora di 4 articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali

Le novelle sono innanzitutto riferite alla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, stabilendo nuovi termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi. Ulteriori innovazioni riguardano la nomina di un nuovo comitato di esperti, deputati allo svolgimento dell'istruttoria sulle predette modifiche e la limitazione dell'applicazione della disciplina vigente, riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali prevista per i proprietari dei siti oggetto di bonifica, ai beni, alle aziende e ai rami d'azienda oggetto del trasferimento. In base al quadro delle norme introdotte dal decreto-legge in esame, al nuovo comitato di esperti è affidato lo svolgimento dell'istruttoria relativamente alla valutazione delle modifiche e/o integrazioni del piano proposte nell'ambito delle offerte, nonché all'attuazione delle modifiche medesime, che non viene più affidata al comitato che ha curato la predisposizione del piano ambientale. Il nuovo comma 8.2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede poi l'istituzione, ad invarianza finanziaria, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un coordinamento tra la Regione Puglia, i Ministeri competenti e i Comuni interessati, con l'obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del piano ambientale, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Si prevede la riunione di tale coordinamento almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. Il nuovo comma 8.2-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede che la Regione Puglia possa autorizzare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia ad assumere personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del piano ambientale e con procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia stessa. Il comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 disciplina la materia degli oneri reali e privilegi speciali connessi al trasferimento dei siti contaminati oggetto di bonifica. In particolare, si prevede che beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del codice dell'ambiente - in base al quale gli interventi di bonifica dei siti contaminati costituiscono un onere reale sul bene immobile - solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare. La lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 1 in esame consente la proroga del termine ultimo fissato al 30 giugno 2017, per l'attuazione del cosiddetto piano ambientale, ciò su istanza dell'aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA in amministrazione straordinaria, disciplinando la procedura di tale possibile proroga, comunque non oltre i diciotto mesi. La lettera *b)* del citato comma 4 interviene poi sul comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, prevedendo due modifiche a tale disposizione: si prevede che sia estesa anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale; inoltre, a seguito di una modifica apportata alla Camera dei deputati, è stato definito, nella disposizione novellata, l'arco temporale di tale estensione di esclusione, specificando che l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale, per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 ovvero per un periodo ulteriore di proroga non superiore ai diciotto mesi (lettera *b*) n. Si richiama al riguardo quanto stabilito nella sentenza n. 85 del 2013 della Corte costituzionale con la quale quest'ultima ha dichiarato inammissibili nonché prive di fondamento alcune contestazioni mosse alla norma. In particolare la Corte ha respinto l'assunto per il quale il periodo concesso all'impresa costituisca «una vera e propria "cappa" di totale "immunità" dalle norme penali e processuali», anche alla luce dei molteplici controlli cui la stessa è sottoposta. Nel corso dell'esame presso la Camera è stato introdotto anche il nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 1, che novella l'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, cui viene aggiunta una nuova previsione, in base alla quale qualora i rifiuti oggetto di recupero siano siano utilizzati fuori dagli stabilimenti ILVA, si applica il *test* di cessione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998. L'originaria formulazione del citato articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2015, prevedeva la conformità a tali *test* unicamente dei residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto, ai fini di un loro riutilizzo per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie o per riempimenti e recuperi ambientali. Mi preme, infine, menzionare l'articolo 1-*bis*, anch'esso introdotto alla Camera (ulteriore prova del fatto che l'*iter* di conversione è stato aperto a possibili modifiche e migliorie da parte del Parlamento), che introduce l'obbligo di mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società ILVA SpA. Più specificatamente l'articolo in commento prevede che, entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società ILVA SpA. Tale disposizione appare imprescindibile ai fini della piena tutela della salute dei lavoratori che operano all'interno degli stabilimenti e della cittadinanza. Ricordo, inoltre, che la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente, invita l'Unione europea a sviluppare, attuare e sostenere un modello per il censimento e la registrazione dell'amianto in conformità dell'articolo 11 della direttiva n. 148 del 2009. Tra le motivazioni addotte meritano particolare menzione il fatto che le comunità locali non dispongono della necessaria esperienza e presentano gravi lacune per quanto concerne l'esecuzione delle attività di prevenzione e sorveglianza, che spesso sono eccessivamente frammentate, e che, oltre alla dimensione umana connessa a condizioni inadeguate di salute e di sicurezza sul lavoro, il problema del mancato tracciamento e smaltimento dell'amianto si ripercuote anche sull'economia. È indubbio, infatti, che i problemi relativi alla salute sul lavoro, oltre alle implicazioni drammatiche dal punto di vista umano, rappresentano un ostacolo alla crescita e alla competitività, provocando al contempo un aumento sproporzionato delle spese previdenziali. Concludendo vorrei tuttavia richiamare l'attenzione di quest'Aula su una preoccupante discrepanza che, a mio avviso, vige all'interno del *corpus* normativo dell'Unione. Sono del parere che una disciplina frammentata, obsoleta e farraginosa come quella sugli aiuti di stato pregiudichi indirettamente la possibilità di realizzare obiettivi europei imprescindibili come quelli contenuti, ad esempio, nella citata risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013. Il caso dell'ILVA in tal senso è emblematico. Come possono, difatti, realizzarsi obiettivi tanto ambiziosi quanto irrinunciabili come la progressiva eliminazione dell'amianto nel minor tempo possibile su tutto il territorio dell'Unione, o sviluppare procedure di lavoro sicure per i lavoratori che potrebbero trovarsi in presenza di materiali contenenti amianto? Ci troviamo, infatti, di fronte a una normativa sugli aiuti di Stato che, se da una parte, con la lettera *e)* del paragrafo 2 dell'articolo 107 del Trattato

nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione; dall'altra, censurano i 300 milioni di euro concessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, destinati a garantire - cito testualmente - la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione. Colleghi io sono un europeista convinto, e proprio in quanto tale ritengo di vitale importanza, per il destino dell'Unione europea, eliminare storture come questa. Mi permetto, quindi, di cogliere questa occasione per richiedere con forza una tempestiva razionalizzazione e semplificazione della normativa europea e nazionale in materia di elargizione e controllo degli aiuti di Stato, che si concentri in particolare su una revisione del testo dell'articolo 107 del al fine di prevedere un ampliamento sistemico delle esenzioni per i regimi di aiuti destinati a favorire lo sviluppo dell'economia delle Regioni dove il tenore di vita è particolarmente basso, oppure dove si abbia un alto tasso di disoccupazione, nonché del regime di aiuti destinati a sanare

straordinari di necessità e urgenza. Al contempo, l'articolo 70 statuisce, con mirabile sintesi, che le leggi vengono fatte dalle Camere

la straordinaria urgenza, nella migliore delle ipotesi c'è perché si è aspettato fino al giorno di questo decreto-legge per prendere talune misure sull'emergenza che si è verificata quattro anni fa. Quindi, l'urgenza è determinata non dalla situazione ambientale (con tutti i problemi ad essa connessi) dell'ILVA di Taranto, ma è causata semmai dalla cattiva legiferazione che si è fatta con i precedenti dieci con i precedenti dieci decreti-legge, ivi inclusi quelli - anch'essi numerosi - emanati da questo Governo, che non sono riusciti a risolvere il problema. Nella migliore delle ipotesi, non sono riusciti a risolvere il problema perché contenevano anche errori, tanto è vero che questo decreto-legge esordisce

una situazione con gravi difficoltà (profili ambientali, occupazionali e così via) che è ben nota da parecchi anni.

con un decreto-legge, perché il Governo vuole continuare a fare le leggi da solo, perché più le fa da solo più evita di dover sottoporre i suoi provvedimenti ad un giusto e corretto vaglio del Parlamento. Dico un'altra banalità, ma va ricordata perché altre volte sembra che persino noi legislatori ce lo dimentichiamo: il decreto-legge non entra in vigore dopo sessanta giorni dalla conversione in legge, ma entra in vigore subito. Quindi, se ci sono errori, sono sbagliati subito.

passato questo testo in tempi tali per cui delle correzioni ancora si potevano fare; tuttavia la maggioranza ha deciso di non modificarlo in Commissione e

evidentemente non c'è più quella straordinaria necessità ed urgenza che si è verificata quando l'emergenza è stata realmente prodotta.

tutti provvedimenti che non hanno risolto il problema (né quello della popolazione dell'area di Taranto, né quello dei lavoratori del gruppo e neanche quello dei turisti che frequentano quella bella Regione)

Nel merito vediamo che ci sono anche alcuni aspetti sconcertanti: a quattro anni dal prodursi dell'emergenza, nel decreto-legge in esame, che è stato straordinariamente necessario ed urgente presente un provvedimento che concede una proroga di ben diciotto mesi alla scadenza per l'attuazione del piano ambientale sanitario,

si giustificherebbe l'urgenza. No, scadono il 30 giugno 2017, quindi è straordinariamente necessario ed urgente stabilire più di un anno prima (perché il decreto-legge non è stato approvato ieri dal Governo, ma il 9 giugno)

è stata fatta una valutazione totalmente errata dei tempi necessari per risolvere la situazione, o adesso si sta concedendo una proroga totalmente ingiustificata. se la valutazione era stata giusta, allora qualcuno non ha fatto ciò che doveva e si prevede che non lo farà nei prossimi dodici mesi, al punto che bisogna dargli altri diciotto altro punto delicato nel contenuto concerne l'estensione dell'immunità penale e amministrativa per l'esecuzione del predetto piano ambientale non più soltanto al commissario straordinario e ai soggetti da lui delegati (questo sì che è straordinario, (questo sì che è straordinario, ma non straordinariamente necessario ed urgente). Ma questa immunità viene estesa anche all'affittuario e all'acquirente dell'acciaieria. Qui abbiamo un'altra questione degna di qualche commento. commento. È molto curioso: si stabilisce l'immunità di qualcuno; questo vuol dire o che questa immunità è totalmente ingiustificata o che, se è

può darsi che sia vero, ma allora cambiamo quelle leggi, non solo per l'ILVA, perché dopo quattro anni - ripeto - l'urgenza non c'è più (resta l'emergenza perché il problema non è stato risolto). Infine, abbiamo un'altra brutta notizia: il prestito di 300 milioni di euro stanziato dallo Stato in favore dell'ILVA non sarà restituito - come era stato stabilito pochi mesi fa in un altro decreto-legge straordinariamente necessario ed urgente - dalla società vincitrice della gara, ma sarà restituito dall'amministrazione straordinaria dell'attuale Gruppo ILVA, anteponendolo agli altri debiti iscritti alla procedura. In altre parole, i creditori del Gruppo sanno che sono retrocessi di 300 milioni: belle notizie per i creditori e per le imprese che rischiano di fallire, perché dopo quattro anni di intervento lo Stato non riesce neppure a garantire i principali creditori dell'ILVA. Per tali ragioni chiediamo che non si proceda con l'approvazione di questo provvedimento: fate un disegno di legge come si deve

Signora Presidente, che cosa è questo undicesimo decreto-legge n. 98? È sicuramente un dispositivo urgente per il completamento della procedura di cessazione degli stabilimenti ILVA.

le condizioni della sicurezza sul lavoro), della libera concorrenza, delle normative europee e, in ultimo, del Parlamento. Undici decreti-legge in cinque anni. Chiediamoci: viene rispettato il carattere di straordinarietà? Credo proprio di no. È un sistema eccentrico di regole organizzato solo per lo stabilimento ILVA, che pone gravissimi problemi ambientali e sanitari e interferisce palesemente, in maniera reiterata, con la riserva di giurisdizione e con l'obbligatorietà dell'azione penale. Nello specifico, questo decreto-legge estende l'immunità penale e amministrativa non più solo ai commissari e a tutti i loro delegati, ma anche all'affittuario e all'acquirente, soggetti ancora non esistenti, perché

noi ci battemmo molto contro questa estensione dell'immunità, che va oltre al dato amministrativo. L'unico riferimento normativo precedente era quello delle regole fissate al

Invece, nel decreto-legge precedente sono stati allargati anche al penale, senza limiti temporali. Con quello di oggi, allarghiamo non soltanto i limiti

possibili, se non sicuri, sui tempi di attuazione del piano ambientale. Ma cos'è questo piano ambientale? Sono passati quattro anni

2019. Ricordo, però, che noi abbiamo ben 91 morti all'anno soltanto nel rione Tamburi e nel rione Borgo per quanto riguarda la relazione dei CTU della procura di Taranto. Quindi, prorogare l'attuazione di queste prescrizioni di altri diciotto mesi è gravissimo.

il Centro studi salute e ambiente ha dimostrato che il rischio di mortalità in quei giorni aumenta moltissimo, anche se

estesa anche all'acquirente l'impunibilità. Questo comporta che non si potrà ricorrere contro chi inquina. Non si potrà ricorrere, né amministrativamente né penalmente, contro chi continuerà a inquinare. Così viene sottratta al cittadino la possibilità di ricorrere per la tutela dei propri diritti violati. E in tal modo risulta anche leso il principio costituzionale di ragionevolezza, in

Questo per quanto riguarda la salute. Con riferimento alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il prestito di 300 milioni di euro non verrà più restituito da chi acquisirà l'azienda, ma dall'amministrazione straordinaria. Questo rende ancora più precaria la posizione dei creditori, non assistiti dal privilegio, e che sono cioè indietro in lista d'attesa.

ha aperto un'indagine approfondita per valutare se questi aiuti di Stato siano compatibili con la normativa europea

siamo arrivati all'undicesimo decreto‑legge riguardante l'ILVA di Taranto. Credo che già soltanto questo numero basti per giustificare e sostenere la questione pregiudiziale

decreto-legge significa - evidentemente - che non si è stati in grado di affrontare e trovare delle soluzioni ai gravi problemi sanitari, ambientali e anche industriali dell'ILVA di Taranto. È soprattutto, si continua a intervenire con decreti-legge, come questo al nostro esame, profondamente lesivi dei principi costituzionali.

e preoccupanti profili di incompatibilità con la normativa europea in materia ambientale. Dispiace molto che i due relatori non si siano soffermati su questi profili di costituzionalità, esaminati anche in Commissione affari costituzionali.

sta ingenerando grave disorientamento e incertezza per i cittadini, i lavoratori e anche per possibili investitori stranieri.

e degli articoli costituzionali. In particolare, all'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, si modifica in modo grave e palesemente incostituzionale l'articolo 2, comma

connesse all'attuazione dell'AIA e delle misure previste nel piano ambientale. Essa è estesa anche all'affittuario o acquirente, ampliando e rafforzando in maniera inaccettabile disposizioni già evidentemente incostituzionali, che noi avevamo evidenziato più volte come palesemente incostituzionali e avulse - me lo lasci dire, Presidente - da qualsiasi rispetto del principio dello Stato di diritto, con violazione non soltanto del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione,

crea una specie di diritto al disastro ambientale in capo ad alcuni soggetti i cui comportamenti vengono tutelati da una presunzione di liceità. C'è una sorta di diritto a poter violare perennemente la legge. presunzione che, con tutta evidenza, appare ancora più grave e preoccupante per chiunque abbia a mente l'insieme dei problemi complessi, gravi e preoccupanti che, soprattutto sotto il profilo sanitario e ambientale, continuano oggi a tormentare il territorio del sito industriale più importante del Paese, nonostante svariate e molteplici procedure di commissariamento avviate da tempo. Tale disposizione viola i principi di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'articolo 112 della nostra Costituzione, in quanto suscettibile di vincolare il giudice a compiere una valutazione di merito con esclusione della responsabilità penale o amministrativa di alcuni soggetti rispetto ad altri che potrebbero essere coinvolti eventualmente nell'attuazione del piano ambientale, con evidente disparità di trattamento, illogico sul piano penale e amministrativo. Inoltre, l'articolo 1, comma 4,

ad esserci sul territorio e a pesare sulla vita quotidiana delle persone mettendo a repentaglio la salute dei cittadini. È chiaro che ciò comporta una violazione palese

Inoltre, tale disposizione viola palesemente la normativa comunitaria in materia ambientale e, in particolare, con l'articolo 191 del Trattato istitutivo dell'Unione europea

svolta dal Ministero dell'ambiente, in violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione. Non vogliamo tediarvi oltremodo anche sul problema delle violazioni dell'articolo 81 della Costituzione, in relazione alla copertura finanziaria, ma vorremmo segnalarvi invece un'altra violazione palese, con la modifica introdotta dal provvedimento al comma

di una vera e propria regalia nei confronti del privato, di circa 400 milioni di euro, con oneri totalmente a carico della finanza pubblica. È evidente, quindi, che per tutti questi motivi

era più che logico poter pensare ad un intervento attraverso l'uso del decreto‑legge, proprio per cercare di superare l'*impasse* che si era venuto a creare su uno stabilimento così importante per la produzione di acciaio in Italia e soprattutto per quanto riguardava la la tutela del diritto alla salute nella zona di Taranto e in tutta la parte ionico-salentina interessata da questo stabilimento.

soprattutto per quanto riguarda l'uso indebito della decretazione d'urgenza e quindi la violazione continua e sempre più eclatante dei principi costituzionali, così come illustrata illustrata anche nelle precedenti questioni pregiudiziali. E vengo così a quelli che sono i motivi che abbiamo illustrato nella nostra questione pregiudiziale QP4, senza senza entrare più di tanto nel merito, anche se la tentazione - così com'è avvenuto anche per gli altri colleghi - è abbastanza sentita Non ritorno sul fatto che siamo al decimo decreto-legge su questo tema; devo dire però che l'utilizzo della decretazione d'urgenza, secondo principi ormai acquisiti e fissati solennemente dalla Corte costituzionale, deve avvenire a precise condizioni. Tra queste, non si può prevedere la reiterazione, che lede quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione. Il provvedimento, in effetti, stabilizza e prolunga nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento dei nove decreti-legge precedenti; viene quindi meno il criterio dell'urgenza, proprio perché c'è una stabilizzazione sempre più evidente ed eclatante. comporta? Comporta la lesione della certezza del diritto nel rapporto tra i diversi soggetti che si affrontano e che si interfacciano con la questione dello stabilimento ILVA, sia dal punto di vista della tutela dei dei diritti, sia per quanto riguarda la partecipazione alle gare, sia per quanto concerne la popolazione interessata da questo stabilimento. Questa lesione della certezza del diritto comporta poi l'impossibilità di prevedere sia la durata delle norme emanate, sia l'esito finale di queste norme, che vengono continuamente modificate. in particolare eclatanti, visto che facevo riferimento prima alla popolazione, gli effetti sul diritto alla salute, quindi le implicazioni correlate all'articolo 32 della Costituzione. La Corte costituzionale nel 2013, trattando della questione dell'ILVA, aveva fermamente fissato il rigoroso rispetto del cronoprogramma relativo all'AIA. Oggi noi, con questo decreto-legge, vediamo riconosciuti ulteriori diciotto mesi; e questo è sicuramente un qualcosa che collide con i principi costituzionali prima citati. Un'altra considerazione: i decreti-legge a pioggia non hanno portato certamente alcun vantaggio sul piano economico-industriale nell'area tarantina fino ad oggi.

punto di vista socioeconomico in generale. Ma sicuramente tutto ciò ha nuociuto alla tutela dell'ambiente e della salute: non si è realizzato quel bilanciamento, che doveva realizzarsi già con i precedenti decreti, tra l'articolo 41, terzo comma, della Costituzione e gli articoli 9 e 32 sempre della nostra Carta fondamentale.

l'introduzione del comitato degli esperti comporta una violazione del principio del buon andamento, soprattutto per quanto riguarda i concetti dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, come fissati dall'articolo 97 della Costituzione. Peraltro, segnalo che il Ministero dell'ambiente dispone già di strutture all'altezza; bisogna far altresì rilevare che tutto ciò avviene senza alcuna partecipazione della Regione Puglia, che pure è interessata notevolmente dalla questione.

Si è già detto dell'immunità penale ad amministrativa, prima concessa solo al commissario straordinario o a suoi delegati, mentre con questo decreto‑legge viene estesa anche all'acquirente o all'affittuario dello stabilimento. È inutile dire che questa è una violazione palese violazione palese ed evidente dell'articolo 3 e soprattutto dell'articolo 24 della Costituzione, perché si frustra il diritto alla difesa del cittadino, che viene danneggiato dal patto illecito dell'acquirente o dell'affittuario dello stabilimento.

Infine, c'è ancora un'altra violazione, quella dell'articolo 11 della Costituzione, in relazione all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato fondamentale dell'Unione europea. Si parla in questo caso degli aiuti di Stato: 856 milioni che sono già stati oggetto, come ricordato da precedenti colleghi, di indagine da parte della Commissione dell'Unione europea. Tutte queste violazioni, tutti questi evidenti conflitti del decreto‑legge con princìpi costituzionali molto importanti, come il principio di uguaglianza o l'articolo 32 più volte richiamato, ci inducono ad insistere sulla questione pregiudiziale di costituzionalità a fronte di una serie di fallimenti del Governo. Si registra peraltro negli ultimi tempi un *derby* permanente tra il presidente del Consiglio Renzi e il presidente della Regione Puglia Emiliano: un *derby* sterile e

che è senza un orizzonte positivo per quanto riguarda la ripresa della produzione. Si è quindi riusciti a non realizzare nessuna delle premesse dei vari decreti-legge fin qui emanati. Proprio per questo, per l'inconcludenza del Governo, ma soprattutto per i vizi che ho segnalato mio intervento, insistiamo per l'accoglimento della questione pregiudiziale e per deliberare di non procedere all'esame del disegno di legge. Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'ILVA ormai è diventata una storia drammatica che impegna le Aule parlamentari già dalla scorsa legislatura e che il Governo dei tecnici non ha saputo certamente affrontare né risolvere con la dovuta concretezza. Le vicende dell'ILVA hanno soprattutto fatto emergere tutta la fragilità del nostro sistema amministrativo di intervento nelle questioni ambientali La mancanza di chiarezza sui ruoli e sulle competenze degli organi istituzionali interessati al risanamento ambientale e alla riqualificazione del territorio di Taranto ha alimentato una serie di procedimenti penali e amministrativi con controbattute del Governo risultate fino ad oggi molto inefficaci e che hanno creato incertezze che non riguardano soltanto l'ILVA di Taranto ma tutto il sistema industriale italiano. soprattutto permesso l'intervento dell'autorità giudiziaria su questioni che rientrano chiaramente nella sfera delle competenze delle autorità garanti della tutela dell'ambiente e delle direttive comunitarie. Riteniamo che sia stata messa in gioco l'affidabilità e la credibilità del nostro Paese nei confronti degli investitori esteri. I cittadini di Taranto pagano l'irresponsabilità della classe imprenditoriale e industriale del passato e l'irresponsabilità della classe amministrativa locale, che fino ad oggi ha chiuso gli occhi davanti al problema sanitario ed ambientale. I problemi ambientali e sanitari sono ancora più gravi se si pensa che nella stessa situazione di emergenza ambientale e sanitaria di Taranto ci sono anche altri 57 siti di interesse nazionale, per la maggior parte situati a Nord del Paese, verso i quali il Governo deve intervenire con risposte concrete a tutela della salute dei cittadini. Quindi, signor Presidente, dopo più di quattro anni di rinnovo dello stato di emergenza, di continui tentativi da parte del Governo di far fronte alla situazione ambientale ed occupazionale

più della metà di questi decreti-legge in due anni senza ancora risolvere la situazione aziendale e senza ancora proporre una soluzione definitiva e credibile. Eppure, ormai, hanno preso coscienza del fatto che la la cessazione dell'attività dell'ILVA di Taranto comporterebbe un gravissimo pregiudizio, non solo per il tessuto economico e sociale del territorio di Taranto ma anche per gli stabilimenti ad essa collegati e per l'indotto tutto in quanto lo stabilimento di Taranto è l'unico punto dove si lavora l'acciaio l'acciaio a caldo e l'azienda è fornitrice di tutti gli stabilimenti dell'ILVA sul territorio nazionale: Genova, Novi Ligure, Racconigi, Marghera ed altri. Il Governo sta mettendo in gioco un gruppo di 16.200 dipendenti diretti e 10.000 lavoratori dell'indotto, che attualmente versa in una difficile situazione finanziaria a causa dei problemi incontrati nella riscossione dei crediti maturati nei confronti della società ILVA. Secondo il nostro Gruppo, la mancanza di soluzioni credibili ed il protrarsi dello stato di emergenza mette in crisi la stessa affidabilità e credibilità del nostro Paese nei confronti, come dicevo prima, degli investitori esteri. perché conferma l'intervento dello Stato nella gestione dell'impresa del Gruppo ILVA, continuando ad invadere la sfera del privato e prorogando l'amministrazione straordinaria. Il proliferare dei decreti-legge sullo stesso argomento annulla i requisiti di necessità e urgenza. Il decreto-legge permette all'aggiudicatario della gara di presentare domande di autorizzazione di nuovi interventi e di modifica del piano delle misure e delle attività tra l'interesse privato dell'aggiudicatario e l'interesse pubblico per la corretta attuazione delle procedure ambientali. Poi ci sono delle situazioni

e del mare i cui compensi sono posti a carico dell'amministrazione straordinaria dell'ILVA, ossia del soggetto che è il principale interessato al proseguimento dell'attività e successiva cessione del gruppo aziendale; anche in questo caso si profila un confitto di interesse *a)*, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo della restituzione del finanziamento statale, anteponendolo agli altri debiti della procedura;

del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione

commissario della procedura di amministrazione straordinaria, è contrario a quanto disposto dall'articolo 41 della Costituzione, che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata. Continua pertanto a profilarsi una sorta di statalizzazione della società che vede lo Stato invadere la sfera del privato. Infatti, la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza nasce per la ristrutturazione e vendita delle imprese a partecipazione pubblica o operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e forzatamente è stata estesa anche all'ILVA.

mare*. Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi,

La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. È convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il relativo dibattito. Sospendo

per la quale sono state ripartite circa due ore in base a specifiche richieste dei Gruppi. Le dichiarazioni di voto avranno luogo domani mattina a partire dalle ore 9,30. Seguirà la chiama. La Commissione bilancio

*(CoR)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, ancora una fiducia. Abbiamo perduto il conto del davvero imbarazzante che su argomenti così delicati e complessi, durante l'esame dei quali le forze di opposizione peraltro tentato di portare un contributo propositivo e non hanno certamente messo in campo atteggiamenti ostruzionistici, non vi sia la possibilità di approfondire

del nostro Paese, una prospettiva di riscatto che dia risposte adeguate ai temi della

per disciplina mi adeguo, ma non ometto il mio disappunto e il mio senso di disagio.

della procura tarantina per inquinamento ambientale. Credo debba essere interpretato come un monito. La cosa paradossale è che l'urgenza, ormai divenuta cronica, si ripresenta puntuale con lo stesso carico di legittime aspettative, di dolore, di attese deluse e di interrogativi inquietanti. Nove decreti-legge, di cui cinque varati dal Governo Renzi, non hanno fornito sino ad ora risposte convincenti sul piano della sicurezza ambientale, del diritto alla tutela della salute e della occupazione. La cosa più grave cosa più grave è l'assoluta assenza di una visione strategica per il futuro di uno dei territori più belli, della città dei due mari, che rappresenta una punta di diamante

decreto-legge, purtroppo, non ce ne restituisce neanche l'ombra. Non si smentisce la posizione del Governo e 1'atteggiamento di chiusura che ha mantenuto in tutto questo periodo con la sua maggioranza

e di sviluppo del Sud, nel cui contesto la vicenda ILVA si inserisce. Il testo approvato alla Camera e arrivato in quest'Aula conferma queste valutazioni. Anche nell'altro ramo del Parlamento

Lo stesso incremento economico mostra in tutta la sua drammaticità il nervo scoperto dell'attività di monitoraggio da parte dell'Agenzia regionale

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la vicenda ILVA, a quattro anni dalle prime indagini dalla magistratura sull'inquinamento dell'area di Taranto, continua a impegnare per la quinta volta il terzo Governo dei nominati, il Governo Renzi. Sin dall'inizio, con l'Esecutivo dei tecnici guidati da Monti, sono stati assunti dei provvedimenti pasticciati, risultati inefficaci. La questione dell'ILVA ha fatto soprattutto emergere tutta la fragilità del nostro sistema amministrativo in merito a controlli e interventi sulle questioni ambientali di politica industriale. Inadempienze, omissioni, mancanza di chiarezza di ruoli e competenze degli organi istituzionali interessati al risanamento ambientale e alla riqualificazione del territorio di Taranto hanno instaurato una serie di procedimenti penali e amministrativi, provocando tardive e inefficaci reazioni dei Governi, che hanno creato incertezze, che riguardano non solo 1'ILVA di Taranto e gli stabilimenti del gruppo e l'indotto, ma tutto il sistema industriale italiano. L'inerzia iniziale dell'Esecutivo Monti ha soprattutto permesso l'intervento della magistratura su questioni che rientrano chiaramente nella sfera della competenza delle autorità garanti della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Con il sequestro preventivo degli impianti dell'area a caldo del 26 luglio 2012, il polo siderurgico più grande d'Italia e il secondo in Europa è diventato ufficialmente un ecomostro, per responsabilità della proprietà: prima dello Stato, sino al 1995, e poi del privato. Ma è diventato anche simbolo di negligenza, di disprezzo ambientale e di violenza della salute pubblica, anche per responsabilità e complicità dei vari enti territoriali locali e degli organismi di controllo che non hanno vigilato: l'ASL prima e, dal 2003, l'ARPA Puglia. Ancora oggi i cittadini di Taranto pagano l'irresponsabilità della classe imprenditoriale e industriale del passato e, soprattutto, l'irresponsabilità della classe politica e amministrativa locale, che ha chiuso gli occhi sul problema sanitario e ambientale. del tutto evidente che l'unico modo per far fronte all'esigenza di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini è la continuità dell'attività di impresa, perché altrimenti Taranto rischia di diventare una seconda Bagnoli. La chiusura dell'impianto comporterebbe non solo la perdita dei posti di lavoro, ma anche il blocco dell'attuazione delle prescrizioni dell'AIA, con il sito inquinato che resterebbe da bonificare, come già accaduto a Bagnoli, a questo punto con oneri solamente a carico del pubblico. Ecco che questo decimo decreto-legge, varato per mettere una pezza all'inefficacia del precedente, il n. 191 del dicembre 2015, ha lo scopo di assicurare il mantenimento dell'attività dell'ILVA, per tutelare il tessuto socioeconomico e occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto, garantendo allo stesso tempo la tutela ambientale, ma anche degli altri stabilimenti del gruppo collocati al Nord,

i commissari del Gruppo ILVA hanno fallito e non sono riusciti a espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali entro il giugno 2016 ed ecco l'ennesima proroga.

così come il rientro in Italia degli 1,2 miliardi di euro sequestrati alla famiglia Riva, che tutti davano per certi e che invece sono rimasti bloccati in Svizzera per decisione del tribunale elvetico. Entro nel merito delle previsioni del decreto-legge riguardanti l'azienda, che non ci convincono affatto: vengono allungati i tempi della procedura di vendita. Da qui alla fine dell'anno avremo una situazione gestionale che vedrà, da una parte, l'acquirente non ancora nel pieno esercizio delle sue funzioni e, dall'altra, una gestione commissariale che, pur prolungandosi nel tempo, non riuscirà a vedere il completamento del piano ambientale, anch'esso più volte prorogato. L'incertezza che ne deriva rischia di mettere in discussione l'attività dello stabilimento e di far perdere commesse e affidabilità. secondo luogo, dopo la proroga di sei mesi concessa con l'ultimo decreto-legge, ne viene concessa un'altra di diciotto mesi per l'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dello stabilimento; dunque niente conclusione del piano ambientale al 30 giugno 2017, ma a fine 2019. Viene così legittimato un conflitto tra l'interesse privato dell'aggiudicatario e l'interesse pubblico per la corretta attuazione delle prescrizioni ambientali. I lavoratori e i tarantini sottoposti a rischio sanitario ringraziano per il rinvio della completa attuazione delle prescrizioni AIA, che, al di là delle percentuali di facciata che vengono sciorinate, risultano ancora incompiute nella parte più economicamente impegnativa, come si evince analizzando lo stato di attuazione del piano ambientale, aggiornato pochi giorni fa dalla stessa amministrazione

Siamo in ritardo e lontanissimi dal completamento del piano e il suo differimento al 2019 evita solo all'amministrazione straordinaria un bel quattro in pagella. Sulla modifica del piano ambientale contestiamo la scelta del Governo di affidare a un comitato di tre esperti la valutazione delle modifiche proposte dall'offerente. Non ne comprendiamo il motivo, visto che il Ministero dell'ambiente dispone già di una commissione AIA o di istituzioni come l'ISPRA, che potrebbero valutare le proposte in offerta di gara. Ci domandiamo, inoltre, perché questi esperti debbano avere solo una comprovata esperienza in materia ambientale e di impianti siderurgici e non - per esempio - in materia economica, giuridica o sanitaria. terzo elemento critico, che è quello che ci preoccupa di più, è la modifica dell'obbligo della restituzione del prestito ponte di 300 milioni, che era stato concesso per garantire la continuità dell'impresa e superare il periodo di vendita. La restituzione è a carico non più dell'aggiudicatario della procedura di gara, ma dell'amministrazione straordinaria; un bel regalo all'acquirente o affittuario. Questa restituzione del prestito anteposta agli altri debiti della procedura ci preoccupa molto. Perché? Perché rende ancora più incerto il diritto dei creditori del Gruppo ILVA al pagamento dei servizi svolti, riaprendo una lacerazione nei rapporti che era stata ricucita con il decreto n. 1 del 2015, grazie soprattutto all'azione emendativa delle opposizioni, che avevano fatto includere i crediti dei fornitori tra quelli prededucibili. È molto grave rimettere in discussione i pagamenti dovuti alle imprese dell'indotto, ai fornitori e agli autotrasportatori. Ci domandiamo - e se lo domanda anche il Servizio di bilancio del Senato - se, nelle condizioni precarie in cui versa la gestione di impresa, che continua a perdere decine di milioni al mese, ci sia la capacità dell'amministrazione straordinaria di far fronte alla restituzione del finanziamento. Ci interroghiamo, inoltre, sui tempi in cui tale restituzione avrà luogo. Ne vedremo sicuramente delle belle ed è per questo che siamo preoccupati per i creditori, che - lo ricordo - hanno ancora congelati i crediti antecedenti al febbraio 2015. Colleghi, come nei precedenti decreti-legge, ritrovo ancora entusiasmi tra i membri di Governo e maggioranza, ma vi consiglio prudenza. Pesa, infatti, come un macigno la lunga serie di provvedimenti che avete messo in campo in quattro anni per tentare di governare la vicenda ILVA, che fino ad oggi avete dimostrato però di non essere in grado di gestire. Noi ribadiamo quello che è stato il peccato originale, l'errore iniziale su ILVA: la statalizzazione di un'azienda privata. Il commissariamento è stato un atto irresponsabile contro natura perché, nonostante tutte le colpe dei Riva per le mancate misure di mitigazione ambientale e per il grave inquinamento dell'area di Taranto, resta comunque un esproprio di un'azienda privata, peraltro strategica per l'economia del Paese, i cui conti economici non richiedevano una tale misura drastica. Prima di concludere l'intervento, voglio rivolgere un pensiero ai lavoratori del Gruppo ILVA. Le loro proteste dei giorni scorsi sono la prova di come il clima di incertezza sul futuro del siderurgico e la proroga dell'applicazione delle prescrizioni AIA creino tensione e ansia negli stessi lavoratori. Le loro preoccupazioni sul mantenimento del posto di lavoro e sul ruolo che l'ILVA potrà continuare a ricoprire nell'ambito dell'industria siderurgica italiana sono comprensibili. Non sono per nulla chiare le prospettive di un'azienda che, una volta in mano al privato, non potrebbe certo continuare a perdere decine di milioni di euro al mese in un contesto di saturazione, a livello mondiale, del mercato dell'acciaio invaso da quello cinese. Stiamo parlando di oltre 25.000 lavoratori, tra diretti e indiretti dell'indotto, che aspettano nell'incertezza da quattro anni che i Governi di centrosinistra giungano a una soluzione definitiva. Questo decreto-legge non piace alla Lega Nord e a molti altri perché prosegue nella strada dell'incertezza e, soprattutto, riconferma l'intervento dello Stato nella gestione delle imprese del Gruppo ILVA, continuando a invadere la sfera del privato e prorogando l'amministrazione straordinaria. State svendendo ai privati un'azienda privata che avete nazionalizzato, senza averne né i titoli né le capacità. Ci domandiamo chi tra i consulenti di Renzi sia oggi il guru dell'operazione dopo che Guerra se n'è andato. Ci rendiamo conto che avete espropriato la società e i Riva perché erano in ritardo con l'attuazione delle misure del piano ambientale e ora per quello stesso piano concedete agli acquirenti non solo la possibilità di introdurre modifiche sostanziali, ma anche il differimento del termine della realizzazione alla fine del 2019? E non solo: con una norma estendete all'acquirente l'immunità penale e amministrativa già prevista per i commissari straordinari e i loro delegati, alleviando l'acquirente stesso dalle proprie responsabilità non solo con riferimento al passato, ma anche per condotte poste in essere fino all'attuazione del piano ambientale. Per questa è una follia. Termino con un suggerimento. Quando vi renderete conto dell'inefficacia anche di questo decreto-legge e sarete prossimi a varare l'ennesimo, restituite tutto ai Riva con l'undicesimo decreto-legge. Sarà la volta buona perché l'ILVA possa diventare efficiente, non inquinante e redditizia e, dunque, salva e protagonista nel mercato siderurgico italiano e globale.

Signor Presidente, la 5a Commissione si è riunita per esaminare il decreto-legge del 9 giugno 2016, n. 98, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

aveva in animo di votare il parere sul testo e sugli emendamenti domani mattina, ma l'accelerazione del lavoro dell'Assemblea, e in particolare l'apposizione della questione di fiducia, ha cambiato l'ordine dei nostri lavori. In ogni caso, l'esame condotto dalla Commissione ci ha portato a prendere atto delle rassicurazioni fornite dal Governo in ordine alla possibilità di restituzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, ed esprimere quindi un orientamento di parere non ostativo con alcuni presupposti: il comitato di esperti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, al capoverso 8.2 possa effettivamente avvalersi della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli oneri connessi all'aggiornamento della mappatura disposta dell'articolo 1-*bis* dei rifiuti pericolosi o radioattivi presenti all'interno degli stabilimenti della società ILVA SpA, nonché le risorse idonee a farvi fronte, siano in capo ai commissari. Con questi due presupposti,

rappresentanti del Governo, come noto, il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA» meglio conosciuto come il decimo decreto-legge salva ILVA è stato varato dal Consiglio dei ministri il 31 maggio 2016 Il contenuto è semplice e, al contempo, illogico e foriero di ulteriori drammatiche conseguenze: seppure si occupi della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo, assicurando totale centralità alla valutazione del piano ambientale rispetto al fattore economico e industriale delle offerte, prevede uno slittamento generalizzato dei termini. Viene spostato al 30 giugno 2016 il termine per il deposito delle offerte, allontanando, in tal modo, la data ultima per la cessione dell'impianto siderurgico di Taranto. Ma, ancor più incoerente, si palesa l'ulteriore allungamento dei tempi laddove si prevede che le eventuali proposte di modifica del piano ambientale, avanzate dagli offerenti, vengano vagliate preliminarmente da un comitato di esperti nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sostanzialmente, ponendo maggiore attenzione alle "tempistiche tecniche" a cui viene subordinata la cessione, si ha modo di appurarne l'effetto negativo direttamente discendente. Nel provvedimento si legge: «Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti». L'allungamento dei tempi, rispetto alle previsioni, è ancor maggiore se si considera il controllo che verrà svolto dall'Antitrust comunitario. Il piano industriale, o meglio la trattativa, dovrà ottenere il via libera dell'organo comunitario. Pertanto, i tempi di aggiudicazione della fabbrica ionica diverranno effettivamente maturi non prima di dicembre 2016. E ancora, approvato il piano, gli acquirenti avranno tempo fino al 31 dicembre 2019 per realizzarlo, mesi in più rispetto al termine del 30 giugno 2017, già a sua volta prorogato. Sorge spontaneo chiedersi come mai il Governo sia giunto a simili decisioni solamente con l'ultimo decreto-legge salva il decimo dal 2012 ad oggi. Di fatto, tale ulteriore "disposizione urgente" sul percorso di risanamento dell'acciaieria di Taranto non fa che estendere ulteriormente i tempi sia della procedura di cessione dell'ILVA ai privati, sia dei lavoratori per il risanamento ambientale. In tal modo, infatti, si creano le basi oggettive per la chiusura dell'ILVA con un'agonia lunghissima che allontana gli industriali con progetti seri, lascia i lavoratori solo con gli ammortizzatori sociali senza più posti di lavoro e i cittadini con un ambiente avvelenato senza bonifiche. Valga per tutti l'esempio terribile dell'acciaieria di Bagnoli a Napoli. I dati diffusi dagli organi di stampa riportano perdite attuali per l'impianto siderurgico ILVA pari a circa 2 milioni di euro al giorno (nel 2015, si sono registrati 918 milioni di perdite, un dato che va sommato ai 641 milioni del 2014, ai 911 del 2013 e ai 620 del 2012), con un dato mensile che si assesta sui 25 milioni di euro e che, a ogni buon conto, rappresenta una stima del tutto prudenziale. I tempi di conclusione per le operazioni di cessione dell'ILVA, così come descritti, conducono, quale logica conseguenza, a previsioni del tutto negative. Lo slittamento generalizzato dei termini, infatti, comporterà ulteriori perdite, le quali porteranno inevitabilmente alla chiusura degli stabilimenti produttivi, ovvero a un ridimensionamento talmente sensibile da condurre a evidenti criticità per l'intera filiera coinvolta. Non possono, invece, mancare considerazioni positive per la concorrenza tedesca presente nel mercato del siderurgico, la quale occuperà, in tal modo, una porzione di mercato enorme a esclusivo discapito del nostro Paese. Consideriamo che a contendersi l'aggiudicazione del complesso aziendale ILVA parrebbero essere due cordate: la prima guidata dal gruppo Marcegaglia, unitamente ai franco-indiani di ArcelorMittal, e la seconda vede l'alleanza del gruppo Arvedi con Del Vecchio e Cassa depositi e prestiti. Al riguardo, sorgono spontanee determinate considerazioni: l'ipotesi ArcelorMittal, oltre a non rappresentare una cordata italiana in quanto la *joint venture* vedrebbe la partecipazione italiana solo per cento di presenza franco-indiana, non convince data la recente storia della società (nel 2015 con un debito netto pari a 16 miliardi di dollari, e nel 2016, ancora in corso, pari a 12 miliardi di dollari). E ancora, le dichiarazioni dei vicepresidenti, responsabili dell'area fusioni e acquisizioni di ArcelorMittal, Ondra Otradovec e Geert Van Poelvoorde, circa i piani della multinazionale sull'ILVA non fanno presagire nulla di positivo sul futuro lavorativo dei dipendenti. Al riguardo, infatti, costoro descrivono una nuova acciaieria con una produzione di 6 milioni di tonnellate all'anno, con tre altiforni. Successivamente, potrebbero aumentare i livelli produttivi sulla base di un'adeguata domanda e di una congiuntura economica favorevole. In altri termini, il livello occupazionale dovrà essere proporzionato ai livelli produttivi. Tali decisioni, però, comportano ricadute inevitabili sui livelli occupazionali. Sul punto, occorre considerare come una produzione basata su simili cifre comporterà inevitabili ricadute; tra prepensionamenti, ricollocazioni e scivoloni vari con la nuova conformazione dello stabilimento si potrebbe giungere a circa 2.500-3.000 lavoratori in esubero nonostante il Governo stimi, al riguardo, circa un migliaio di unità. Con buone probabilità, tale ultima previsione rappresenta un eccesso di ottimismo, dato che nell'area a caldo sono, infatti, impiegati circa i due terzi dei lavoratori dello stabilimento ILVA. Le precedenti acquisizioni di importanti aziende siderurgiche in Italia non hanno certo brillato per sviluppo, investimenti e nuovi posti di lavoro; anzi, basti vedere il caso di Magona a Livorno in cui da anni si utilizzano ammortizzatori sociali. Il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, ha più volte dichiarato come l'ILVA rappresenti un interesse nazionale in quanto azienda che ha effetti su tutta la catena produttiva italiana. Al contempo, però, il Ministro non ha chiarito in che modo verrà garantita, almeno prevalentemente, la presenza italiana; così come, rispetto ai tempi di attuazione del piano industriale, ha confermato e ribadito quelli previsti dal decimo decreto-legge salva ILVA: *in primis* la presentazione delle cordate alla fine del mese di giugno 2016, poi la presentazione del piano ambientale, che verrà analizzato in centoventi

Persistono le criticità connesse allo stabilimento ILVA di Taranto, con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli impianti, ai risvolti ambientali, al mantenimento degli assetti produttivi e dei livelli occupazionali, ivi compresi i lavoratori dell'indotto, costretti da tempo a subire un grave danno salariale. Le vicende giudiziarie, il processo in corso per il presunto disastro ambientale e la condanna di Fabio Riva per truffa ai danni dello Stato per 100 milioni di euro realizzata attraverso l'ottenimento di contributi pubblici,

purtroppo, a una lenta agonia (facendo, però, la felicità dei concorrenti). Un esempio del dramma che ci si prepara lo abbiamo già visto con Bagnoli. quindi, che il Ministro si assuma la responsabilità delle decisioni prese proprio in termini temporali. Allo stesso tempo, il nostro voto come Italia dei Valori è legato

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'oggi siamo ad adottare l'undicesimo decreto-legge su un tema delicatissimo. Ho detto l'undicesimo, ma in realtà sono molti di più quelli che, direttamente o indirettamente, hanno interessato l'ILVA. Da tutto ciò emerge limpido un dato: il Governo non è in grado di individuare soluzioni definitive per il polo industriale di Taranto. Si sta intervenendo - lo sottolineo - con piccole e limitate operazioni che non parlano quasi mai di strategia, di futuro. Il Governo, inoltre, ha un altro grande difetto in questa annosa vicenda: non ascolta chi vive sul territorio tarantino e potrebbe, quindi, fornire proposte concrete a questioni complesse. In tutto ciò, nel frattempo, le cose continuano a diventare sempre più difficili. Cittadini e lavoratori di Taranto meritano un altro metodo; anzi, direi un'altra politica, nel senso più autentico della parola. Per carità - lo abbiamo già detto - la vicenda è spinosa e complessa. Bisogna legare due interessi di enorme valore: tutela ambientale e occupazione. Non si fa però nulla di reale, nemmeno per iniziare a lavorare su questo fronte. Noi Conservatori e Riformisti, unitamente a quanto sostiene l'onorevole Raffaele Fitto, riteniamo che questo ennesimo decreto-legge sia solo un'altra pezza che non risolve alcunché. È solo il modo per guadagnare inutilmente tempo a danno della città di Taranto e della sua Provincia. L'ILVA è una questione nazionale: non è tarantina né pugliese né meridionale, ormai stanchi di ripeterlo. Questo Governo, però, fa finta di non saperlo o di non volerlo sapere. Per tale motivo, agisce con operazioni più simili a *spot* pubblicitari che a concreti piani di intervento. Se così non è, ci dica concretamente che cosa ha in mente per risolvere l'emergenza sanitaria e ambientale dell'area. Ci dica come e cosa vuole fare per mantenere vivo e moderno questo grande stabilimento centrale per l'Italia e l'Europa. Andiamo al merito del decreto-legge di oggi. Stiamo per convertire un testo che interviene nuovamente sulla procedura di cessione dell'ILVA a soggetti terzi. Si parla, inoltre, di guidare la delicata fase di passaggio con un'adeguata tutela dell'ambiente e della popolazione. Io, però, vorrei sottolineare tre punti. Per quanto riguarda il primo, il decreto-legge prevede per l'amministrazione straordinaria del Gruppo l'obbligo di restituire degli importi erogati dallo Stato. il decreto-legge prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un coordinamento tra la Regione Puglia e altre amministrazioni statali per favorire lo scambio di informazioni sull'attuazione del cosiddetto piano ambientale. Terzo punto: entro fine anno, i commissari straordinari devono trasmettere al Ministero dell'ambiente la mappatura, aggiornata al giugno 2016, dei rifiuti pericolosi e del materiale contenente amianto presenti negli impianti ILVA. Sono tutte questioni che rischiano di ampliare il problema. Cosa accadrà, ad esempio, se gli importi di cui si è detto poco fa non saranno restituiti dai commissari? Nulla si dice nel provvedimento.

per il settore industriale, già gravato da costi energetici esorbitanti. Ma vi è di più. Anche l'Europa è intervenuta pesantemente sulla questione ILVA. Vorrei, infatti, che la Commissione europea ha deciso di andare avanti nell'indagine sugli aiuti di Stato concessi dal Governo al polo tarantino, aspetti a dir poco spinosi che non vengono assolutamente affrontati dal decreto-legge che stiamo per affrontare. Per tali motivi, in conclusione, a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti, dichiaro la nostra forte critica verso un provvedimento che ha misure inefficaci che non affrontano in nessun caso i problemi seri del polo industriale tarantino e di cittadini e imprese dell'area. Signor Presidente, siamo qui a parlare dell'ILVA, del decimo decreto-legge ILVA: dieci decreti-legge più alcuni aggiustamenti inseriti nella legge di stabilità. Questo ennesimo provvedimento credo si possa considerare un sintomo. Mi spiego meglio: è il sintomo che la vostra politica economica, basata su questo tipo di politica industriale, non funziona più. Non solo non funziona più, ma è totalmente fallimentare. Le cose sconvolgenti e sconsiderate sono due. La prima è continuare a far finta che tutto andrà bene e che la vostra visione sia non solo l'unica possibile, ma anche quella giusta. La seconda è che applicate la stessa metodologia anche per risolvere la questione banche, ormai diventato problema del sistema bancario. Solo che in questo caso, per risolvere il problema del sistema bancario, avete intenzione di utilizzare il risparmio postale degli italiani, sempre attraverso Cassa depositi e prestiti. Il risparmio postale degli italiani è ormai l'unica cassa che tiene in piedi il Paese Italia e voi avete intenzione di utilizzarlo per prestare garanzia al sistema bancario. Quella che avete intenzione Quella che avete intenzione di fare, per lo più con soldi non vostri, la trovo veramente una manovra molto azzardata, perché il risparmio postale è l'unica ancora di salvezza per il Paese e voi fate una scommessa che non sappiamo come andrà a finire.

gli imprenditori si suicidano per la disperazione; i risparmiatori si suicidano perché sono stati truffati e ora volete impegnare i soldi dei pensionati. Io capisco che il Fondo monetario internazionale affermi che la longevità dei Paesi mediterranei sarà un problema di bilancio,

e anche l'ILVA in questo caso, ma i pensionati dovranno accendere un mutuo per integrare la pensione e sopravvivere. Sempre seguendo il Fondo monetario internazionale (che mai avrei pensato di citare), vorrei capire dove sono i piani d'emergenza nel caso in cui i mercati finanziari ormai globali imploderanno su loro stessi. Di certo non è pensabile da un giorno all'altro cambiare il sistema, ma credo che ormai non sia più rimandabile. Serve un progetto chiaro e a lungo termine, basato su paradigmi del tutto diversi, che preveda tempi di transizione tra vecchio e nuovo, con tappe ben precise e definite. Con la visione politica che voi portate avanti con una determinazione incomprensibile, non solo non si vede un sereno futuro, ma quel futuro è già tutto ipotecato. Ricordo, infatti, che son rimaste clausole di salvaguardia per 15,133 milioni di euro per quanto riguarda l'anno 2017, per 19.571 milioni per il 2018 e per 19.571 milioni per il 2019: un totale di clausole di salvaguardia per 55 miliardi di euro (se vogliamo essere precisi, 54.375 milioni). Inoltre, ogni anno sono previsti, in media, 5 miliardi di interessi per i derivati che sempre voi avete stipulato, su cui c'è sempre di più un segreto e non si può sapere cosa stia succedendo. Quindi, sui prossimi tre anni pesano già 70 miliardi di euro, senza avere nemmeno iniziato a pensare alle esigenze reali. Questo vuol dire che, per fare le vecchie finanziarie, avete già ipotecato i prossimi anni, il 2017, il 2018 e il 2019, e ancora non avete risolto nulla e non avete neppure un obiettivo. Continuate a mettere toppe su toppe, come su una vecchia strada, ma sappiate che in fondo a quella strada ci aspetta il baratro, per colpa vostra.

abbiamo rilievi costituzionali sugli articoli che riguardano la tutela della salute, la tutela ambientale e la sicurezza, la libertà e la dignità umana; abbiamo rilievi in materia ambientale da parte dell'Unione europea e gravissima emergenza industriale sanitaria e ambientale, che continua ad essere affrontata con provvedimenti d'urgenza che sino ad oggi hanno dimostrato tutti i loro limiti Il metodo e la filosofia degli interventi del Governo sul drammatico caso dell'ILVA non hanno, infatti, ancora prodotto risultati concreti per la salvezza dell'azienda, né per il futuro delle sue famiglie, dei dipendenti e delle numerose imprese dell'indotto e dei loro lavoratori. L'adozione di questo ennesimo decreto-legge non si giustifica alla luce del fatto che l'intervento statale è idoneo solo se temporaneo e transitorio. Spero che il Governo si interroghi sugli effetti dei tanti decreti d'urgenza e sulle cause probabili della loro inefficacia. L'ILVA è sottoposta alla gestione statale fin dal 2013, prima attraverso il commissariamento per ragioni ambientali, poi attraverso l'amministrazione straordinaria con la nomina dei commissari straordinari. In pratica, parliamo di un'impresa che è stata sostanzialmente espropriata, ma in tutti gli interventi non c'è mai stato alcun riferimento al lungo periodo, né si è intravisto un orizzonte temporale al di là di qualche mese,

quello della necessità di un piano industriale è un aspetto fondamentale per non trasformare ogni provvedimento per l'ILVA in una beffa per il territorio, per i lavoratori già stremati da un'attività che non può più

finora - ahimè - negoziati, accordi e normativa a supporto non si sono dimostrati all'altezza della situazione. governativa non si è dimostrata in grado di gestire una vicenda che riguarda non una semplice impresa, ma l'impresa siderurgica che gestisce il più importante polo produttivo dell'acciaio in Europa, rappresentando una componente fondamentale di tutta la siderurgia del nostro Paese. Non disconosciamo la complessità della vicenda, ma un Esecutivo all'altezza della situazione avrebbe avuto un altro passo, un altro approccio strategico, un'altra visione delle politiche industriali italiane. Le continue proroghe dei termini, poi, determinano un'evidente confusione anche nei potenziali acquirenti, ben coscienti del rischio cui sono sottoposte queste disposizioni, nonché tutte quelle intervenute in precedenza. E a proposito dei gruppi finanziari e/o industriali interessati all'ILVA, nulla di serio è stato fatto per risultare convincenti nelle intenzioni del Governo italiano. In ogni caso, lo slittamento del termine per l'attuazione del piano di risanamento ambientale è da considerarsi una vera e propria follia, soprattutto se a questa disposizione si aggiunge l'incertezza sulle responsabilità penali e amministrative dello stesso risanamento, nel caso in cui un gruppo industriale subentri nella gestione dell'impresa. Detto questo, rimane il problema dei problemi, che questo decreto-legge non affronta per niente e che costituisce il tema centrale. I cittadini dì Taranto chiedono che venga verificato quanto il tasso di inquinamento provocato abbia inciso direttamente sul danno sanitario che molti tarantini e pugliesi vivono sulla propria pelle e su quella dei propri familiari, deceduti per patologie tumorali o cardiorespiratorie. Questo decreto-legge non affronta, in buona sostanza, il problema, ed è il motivo principale per cui, ancora una volta, abbiamo, come Conservatori e Riformisti, provato a proporre delle modifiche che in Commissione sono rimaste inascoltate. Sarà la volta buona? I precedenti non depongono bene. Per questo mi associo, modestamente, nel dare voce alla comunità pensante tarantina e meridionale, che manifesta delusione

Presidente, ho poche cose da dire, perché si è detto tutto sulla retorica di questi decreti-legge sull'ILVA.

che si alzano in piedi e drizzano la schiena nel momento in cui noi parliamo di sostegno alle piccole imprese o di reddito di cittadinanza e si scandalizzino perché dicono che siamo statalisti e assistenzialisti. Voi, invece, siete quelli vogliono fare, che vogliono andare avanti, che non piagnucolano e non stanno lì a lamentarsi. Questo lo dice il vostro *Premier*. È strano ed è molto incoerente. Poi state lì a parlare di occupazione e di posti di lavoro, argomenti che non conoscete.

a fare una gita a Taranto e magari ad affittare o comprare un appartamento nel rione Tamburi. Potrebbe magari cogliere l'occasione di aprire le finestre, nonostante il sindaco abbia emanato una delibera in cui chiede ai cittadini di tenere le finestre e le porte chiuse. Taranto, infatti, accade questo. Soltanto la settimana scorsa il sindaco ha emanato una delibera con la quale chiede ai cittadini di tenere porte e finestre chiuse. Perché a Taranto non è possibile aprirle le finestre. Nel cuore dell'Europa è meglio tenere le finestre chiuse. Come se questo potesse bastare a non morire di cancro.

avrebbe lottato contro l'Unione europea e li avrebbe salvati. Invece salva di nuovo l'ILVA. Salva di nuovo questa grande industria che in piedi non sa stare, nel vostro silenzio e nella vostra complicità. Di pari a passo a tutto questo, il nostro Sud si vede ancora depauperato e impoverito dai nuovi gasdotti, da Cerano, da una centrale a carbone che ammazza anche a Brindisi. E tutto viene ingigantito e aggravato dall'ILVA, perché i venti non arrivano solo sulle finestre e sulle porte di Taranto

nuovo, quelli che vanno incontro a chi vuole fare impresa, a chi finalmente ce la fa da solo e non si lamenta. L'ILVA non è quella! Fatela chiudere!

ispirandosi al ragionevole bilanciamento di questi diritti fondamentali. Questo percorso è stato avallato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 2013, che ha rigettato e dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla procura di Taranto con riferimento al secondo dei decreti-legge di questa serie, individuando proprio nell'azione del Governo questo ragionevole bilanciamento tra interessi e valori tutti primari. Infatti, nell'ambito

indicazioni che ci vengono dalla Commissione europea e, dall'altro, per agevolare la conclusione di questo percorso con la cessione del complesso industriale a un gruppo che riprenda a pieno ritmo l'attività produttiva e garantisca i livelli i livelli occupazionali. Al primo obiettivo risponde lo spostamento sull'amministrazione straordinaria dell'onere del rimborso dei 300 milioni di prestito; al secondo obiettivo risponde, per esempio, la possibilità per gli offerenti di proporre modifiche al piano ambientale. È vero che il piano ambientale è stato adeguato alle migliori tecniche disponibili con quattro anni di anticipo: entrato in vigore in tutta Europa a metà del 2016, il piano ambientale è stato adeguato a quelle tecniche già nel 2012. Siamo nell'ambito della tecnica, della scienza e della tecnologia ed è possibile

prima dell'individuazione dell'aggiudicatario. Risponde a questa esigenza anche l'aspetto, da tutti giudicato scabroso, dell'esenzione ed esclusione della responsabilità penale o amministrativa per atti che siano

non determini ulteriori stop al processo di risanamento di quell'area e alla ripresa dell'attività produttiva. Concludo dicendo che il Governo fa bene a difendere questo settore e a puntare i piedi in Europa, chiedendo di rivedere le norme sugli aiuti di Stato alla siderurgia. Mi fa specie che chi ogni giorno grida contro quest'Europa dei vincoli, dell'ottusità e dei limiti, poi richiami le procedure procedure di infrazione che l'Unione europea attiva nei nostri confronti quando si tratta di difendere un interesse nazionale. dell'acciaio e della siderurgia c'è l'interesse di altri Paesi che premono sull'Europa perché Taranto chiuda, ma è interesse dell'Italia che Taranto rimanga aperta. Signor Presidente, come noto a tutti, il decreto-legge interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, relativamente alla modifica e all'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, nonché ai diritti e agli obblighi degli acquirenti o degli affittuari del complesso aziendale. A partire dal 2012 questo è l'undicesimo decreto-legge che, in un modo o nell'altro, tenta di affrontare i problemi dell'ILVA. Questo nuovo intervento prevede una serie di modifiche all'impianto normativo adottato per la cessione dell'azienda e dei suoi *asset*. Lo stabilimento, che oggi conta ancora 12.000 dipendenti, registra una perdita di 2,5 milioni di euro al giorno (come evidenziato dal «Corriere della Sera») e da tre anni non pubblica un bilancio consultabile. L'ultimo è di tre anni fa. Lo Stato, pur di cederlo, di cederlo, ha di nuovo messo mano alla normativa. L'obiettivo dichiarato di alcuni decreti dell'Esecutivo era quello di sottrarre la gestione dell'ILVA al gruppo Riva per darlo, allo Stato, il quale, secondo il Presidente del Consiglio, l'avrebbe dovuta trasformare in un esempio a norma. Non ci si è riusciti e, quindi, si vuole vendere la fabbrica senza aver risolto il nodo della messa a norma, incentivando il privato fino al punto di liberarlo da ogni problema con l'immunità penale, la possibilità di scrivere il piano ambientale senza prescrizioni pubbliche (seppur con un presunto controllo preventivo di esperti) e prevedendo il fatto che, anche nel caso in cui il piano «validato» non dovesse essere realizzato, ci possano essere possibilità di proroghe. In particolare, è previsto che la restituzione del prestito di 300 milioni di euro (per il quale è stata già estesa un'indagine della Commissione europea) non sia più a carico dell'acquirente, ma della stessa ILVA. Poi si disciplina il subprocedimento che si dovrebbe aprire dopo la presentazione delle offerte. Infatti, durante questa fase, l'offerente presenta il piano ambientale al comitato di esperti, con le modifiche a quello già approvato. Il comitato di esperti entro centoventi giorni deve formulare le proprie osservazioni e le proposte di modifica. Questa misura si configura come una vera e propria inaccettabile contrattazione tra l'offerente e il comitato di nomina ministeriale. Come ho già detto in Commissione, come si fa a dire «sì» se a chi acquista o affitta ILVA sarà data l'immunità penale? non sarà obbligato, in maniera certa, a fare le bonifiche? Se potrà cambiare il piano ambientale e sanitario e, se, per ultimo, avrà un'ulteriore proroga di diciotto mesi per la realizzazione delle prescrizioni ambientali strettamente connesse alla salute dei lavoratori e della popolazione tarantina? Come si fa a dire «sì» ad un decreto-legge che estende l'immunità penale, già prevista per i commissari straordinari ILVA, per le condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale, anche agli acquirenti ed affittuari dell'azienda? Tale prescrizione si ritrova all'articolo 1, comma 4, Significherebbe di fatto dire «sì» ad un'assurdità, ad un diritto da «fantascienza». Non dimentichiamo che il comitato Legamjonici ha promosso, nel 2013, il primo ricorso collettivo alla Corte europea dei diritti umani, seguito da un altro ricorso del 2015, presentato da altri ricorrenti. L'Italia è oggi sotto processo ed ha l'obbligo di presentare le proprie osservazioni entro il 30 settembre prossimo, in seguito all'ottenimento anche qui di una proroga. di una proroga. Dovremmo tutti qua dentro dire forte che non sono le deroghe, gli strappi alla legalità e le eccezioni le strade per un buon rapporto tra industria, ambiente e salute. Roberto Della Seta, ecologista, già presidente di Legambiente e senatore del PD, oggi fondatore di Green Italia, ha scritto dietro quasi tutti i decreti salva ILVA vi è una stessa "filosofìa": ILVA va tenuta in vita ad ogni costo, perché dà lavoro a migliaia di persone e perché l'acciaio è una produzione strategica. Va tenuta in vita anche a costo di ridimensionare un po' le garanzie a tutela della salute e dell'ambiente. In realtà, reputo - e reputiamo tutti - vero l'esatto contrario: produrre acciaio, come ogni altro manufatto, infischiandosene delle leggi e della salute non è "moderno", non è "economico" e va contro ogni logica di mercato. Che l'ILVA fosse o potesse diventare un problema lo si era capito sin dagli anni Settanta. Dopo quarant'anni, non mi sembra che ci sia una grossa differenza. In un cablogramma *top secret* pubblicato da Wikileaks, si spiega già il fallimento delle politiche locali e nazionali sulla città di Taranto. Questo scrivevano gli americani: «Taranto è una (...) città dell'acciaio nel vecchio meridione d'Italia. È considerata un banco di prova in Italia per l'industria di base ad alta intensità di capitale come mezzo per stimolare lo sviluppo economico nel Sud Italia. La maggior parte degli osservatori ritiene che l'esperimento non abbia avuto successo». Questo veniva scritto circa quaranta anni fa. E ancora: «Taranto è afflitta da diversi problemi: è una città dove è presente un unico gruppo industriale, senza un'adeguata pianificazione locale e nazionale, con un'amministrazione locale inefficiente e una classe politica scadente e spesso corrotta. A questi motivi di sofferenza si aggiunge la prospettiva di una crescente disoccupazione a causa della fine del *boom* edilizio locale e della sovrapproduzione mondiale dell'acciaio». Ancora, sempre secondo questo cablogramma: «La prosperità e l'occupazione pressoché a tempo pieno a Taranto non hanno prodotto il grande miglioramento della qualità della vita che ci si attendeva. Certamente non hanno stimolato la crescita economica secondaria che molti si aspettavano. Una *leadership* locale inadeguata su tutti i fronti, insieme ad alcune scelte politiche sbagliate (e la povertà di ciò che è stato portato a termine) hanno contribuito a questi scoraggianti risultati. La situazione di Taranto verrà citata come un'ulteriore ragione - in aggiunta alla capacità eccedente - per opporsi alla costruzione di un quinto stabilimento siderurgico italiano a Gioia Tauro in Calabria». Questo scrivevano gli americani: poi sappiamo come è andata a finire con Gioia Tauro, cosi come sappiamo, ed è sotto gli occhi di tutti, che non si sono prodotti grandi miglioramenti nella qualità della vita, come ci si attendeva: anzi, tutt'altro. Infine, muovo una ulteriore critica esplicita al Governo. Come si fa, solo per far vedere che il Governo è buono e disponibile (nella fattispecie, mi riferisco alla sottosegretaria Bellanova), ad accogliere, con parere favorevole, un ordine del giorno alla Camera

questa Europa, così come è strutturata, sia destinata a fallire, soprattutto per i sacrifici che impone ai suoi cittadini e ai suoi lavoratori. Si tratta infatti di un'Unione europea basata soprattutto sul profitto e lo scambio di merci; un'Europa votata

anche solo pensare che uno Stato non possa erogare aiuti pubblici per la ristrutturazione di imprese in difficoltà, in particolare quando si tratta di imprese che dovrebbero rappresentare un fiore all'occhiello, un interesse strategico nazionale da proteggere e preservare a qualsiasi costo: imprese la cui demolizione implicherebbe la distruzione non solo di una città o di una singola Regione, ma dell'intero Stato. Mi riferisco alla lettera inviataci

Una demolizione che presuppone la perdita di migliaia di posti di lavoro e di vite umane. Mi domando come si possa parlare di competitività degli Stati europei, quando gli stessi non viaggiano alla stessa velocità. Secondo il mio parere, si può parlare di una giusta e sana competitività solo quando i concorrenti hanno fin dalla partenza le stesse opportunità e risorse; altrimenti, si rischia che a vincere siano sempre gli stessi, quelli che partono già avvantaggiati. Ma, al di là di questo, non trovo sia giusto su nessun piano che lo Stato non possa farsi carico della ristrutturazione dell'ILVA, che al contrario dovrebbe essere nazionalizzata con una gestione messa a punto dagli operai, pensando a tutti quei lavoratori che nel corso degli anni si sono ammalati e sono morti in nome del profitto dei soliti. Perché, se ad uno Stato non permetti di salvare le sue eccellenze, in particolare in un periodo di profonda recessione, si rischia che l'intera Italia diventi un'area di crisi industriale e sprofondi verso perdite irreversibili. Perché non concedere ad uno Stato la possibilità di autoregolarsi e di gestire le problematiche che solo lo stesso può conoscere alla perfezione fa completamente venir meno il concetto di sovranità. E, senza sovranità, di che Stato stiamo parlando? Se poi lo scopo è quello di far sì che un altro pezzo della nostra storia industriale venga svenduto, allora questa fantomatica Unione dovrebbe dirlo subito, chiaro e tondo. Com'è avvenuto con Italcementi, a discapito prima di tutto dei lavoratori. E invece ecco l'ennesimo decreto-legge nostrano, che vorrebbe gestire una vicenda così importante e delicata con superficialità e senza un piano concreto proiettato sul lungo periodo. Zero visione prospettica e miliardi di euro spesi per rattoppare qua e là, in caso di di primo bisogno, senza la benché minima pianificazione. L'Esecutivo, piuttosto che tutelare i cittadini dopo anni di disastri ambientali che sono andati a minare la salute e il lavoro di una grossa fetta della popolazione, cerca di porre rimedio

per giunta estesa anche ai futuri acquirenti e ai loro delegati, come un incentivo a non dover rendere conto dei risultati dell'attività che si andrà a svolgere, senza alcuna effettiva garanzia per i livelli occupazionali. 300 milioni di euro non saranno più messi in carico al soggetto che subentrerà, ma tali costi andranno nuovamente a ricadere sullo Stato e di conseguenza sui cittadini, che si troveranno a pagare l'inefficienza di una gestione commissariale. modo, l'autorizzazione integrata ambientale potrà essere modificata a proprio piacimento da chi gestirà le sorti dell'azienda. E ad oggi non sono state attuate misure idonee atte

Ma andate a dirlo a tutti i familiari delle persone che hanno perso affetti, sostentamento e ingenti risorse per le cure mediche. D'altronde, qui viene in soccorso il principio di matrice internazionale secondo cui "chi inquina paga", che si concretizza nel fatto che che non paghi nessuno o che, per maggiori profitti, spesso convenga continuare ad inquinare e mettere in conto qualche soldino di multa. Così le soluzioni sembrano essere sempre scaricate sulle spalle dei cittadini e dei lavoratori, laddove vige la legge del massimo profitto e dove la messa in sicurezza del territorio diviene soltanto un inutile orpello.

è passato un anno da quando, con la Commissione di inchiesta sugli infortuni e sulle malattie professionali, ci siamo recati all'ILVA di Taranto. Devo dire che nulla è cambiato, se non in peggio. Quello che era emerso ascoltando i lavoratori, i loro rappresentanti, le associazioni dei malati e di chi non c'è più e gli organi competenti locali era chiarissimo: lavoro sì, ma lavoro dignitoso e non a discapito della salute dei lavoratori e della gente del territorio. A me questo è sembrato di capire, e chi mi vuole smentire lo faccia. Hanno chiesto di essere tutelati dalle istituzioni e quindi di non essere abbandonati dallo Stato e dalla politica, perché il prezzo che hanno pagato in quel territorio, e che ancora pagano, è insopportabile sul versante della sicurezza e della salute. Invece, ancora una volta, non si ascolta il territorio e non si ascolta la gente. Siamo praticamente all'undicesimo provvedimento d'urgenza: è chiaro quindi che gli altri dieci hanno miseramente fallito. È un nuovo provvedimento - si fa per dire, naturalmente - in linea con i precedenti, cioè vuoto, che non da nessuna risposta né ai lavoratori né al territorio. Infatti, questo provvedimento prevede che i potenziali acquirenti mettano a punto un piano ambientale che sarà poi valutato in centoventi giorni da tre esperti: si ritorna indietro, come se nulla fosse successo in questi anni, come se le richieste dei lavoratori e dei cittadini di quel territorio nulla abbiano a che fare con la verità. Eppure le richieste avanzate alla nostra Commissione erano chiare e fattibili. La prima: copertura dei parchi primari; la seconda: aspirazioni di polvere GRF (gestione rottami ferrosi); la terza: sistema Proven alle batterie di cokeria, che è un sistema brevettato d'avanguardia per il controllo della pressione del forno; la copertura integrale dei nastri trasportatori (oggi siamo circa al 65 per cento). Ma la richiesta che è venuta ancora più forte e chiara da tutti gli organi che abbiamo ascoltato era di potenziare gli organi preposti al controllo sulla sicurezza. Io ho fatto dei passaggi, perché ho molti contatti lì, e non mi risulta che questo sia stato fatto; anzi, addirittura mi viene detto da fonti molto attendibili che non hanno neppure i mezzi

Mi hanno anche detto che Taranto ha bisogno di maggiori attenzioni e risorse dal punto di vista della prevenzione e dell'offerta sanitaria, vista la criticità in cui versa, ma questi provvedimenti necessari non sono nemmeno lontanamente previsti in questo vostro nuovo provvedimento.

Addirittura, e lo sanno tutti comprese le pietre, con questo provvedimento non si vincolano neppure i futuri imprenditori, se ci saranno, a garantire i livelli occupazionali:

Un altro problema che i lavoratori, le associazioni e i sindacati hanno sollevato riguarda, la situazione di emergenza che grava sulle migliaia di lavoratori dell'indotto,

il lavoro ci deve essere ma a patto che non si pretenda la sicurezza. È veramente allucinante! È veramente allucinante! Io credo che sia una cosa non degna di questo Paese, una cosa che offende che offende questo Paese tutto e offende quel territorio che ha già pagato un prezzo veramente altissimo da questo punto di vista.

quando interviene la magistratura su temi inerenti al lavoro e alla sicurezza sul lavoro, quando la magistratura è costretta ad intervenire su questi temi, vuol dire che la politica ha fallito

26.999 ricoveri, 3.857 all'anno. Considerando solo i quartieri di Tamburi e di Borgo, che sono più vicini allo stabilimento, abbiamo 637 morti, 91 morti all'anno 4.536 ricoveri, 648 all'anno. Questi sono i dati della perizia epidemiologica dei periti di parte della procura di Taranto. Di questo parliamo quando parliamo di ILVA. Sono esiti per cui esiste e viene dichiarata la forte evidenza scientifica di un possibile danno attribuibile proprio allo stabilimento. Non voglio più parlare solo con le nostre parole o con le parole degli ambientalisti. Ci terrei riportare e leggere testualmente anche i pareri di altri enti o soggetti,

La relazione sintetica dell'ARPA Puglia dice: «Le criticità ambientali connesse all'attuale attività dell'ILVA, di cui agli allegati, mostrano come già allo stato attuale, a causa del non completamento delle prescrizioni AIA e comunque della loro insufficienza della loro insufficienza a garantire adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria, esista la necessità di una revisione in senso restrittivo dell'attuale AIA e del Piano Ambientale in vigore e comunque la necessità del pieno rispetto delle prescrizioni. Anche la valutazione del danno sanitario, elaborata secondo la legge regionale recepita in AIA, ammessa l'attuazione di tutte le prescrizioni AIA con livelli produttivi superiori ai sei milioni di tonnellate di acciaio annuo» - e tutti i portatori di interesse che sono stati in audizione per il per il precedente decreto-legge ci hanno assicurato che si avrà una produzione sicuramente maggiore a 6 milioni di tonnellate annue - «restituiva un quadro di inaccettabilità del rischio». Queste sono parole dell'ARPA

non solo delle prescrizioni AIA, ma di efficaci misure di contrasto alle criticità evidenziate nel corso dei recenti controlli e monitoraggi, di fatto rappresenta un mantenimento di evidenti livelli di rischio», quelli che sono stati riportati nella perizia di parte della procura.

impermeabilizzazione delle aree in cui avvengono le operazioni di deposito delle scorie non deferrizzate da trattare e delle aree afferenti agli altiforni, nonché quelli di installazione dei filtri a maniche; critica gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti; mancata rimozione delle ingenti quantità di rifiuti stoccati in aree sequestrate e relative operazioni di caratterizzazione delle aree potenzialmente contaminate; cattiva gestione degli eventi anomali, malfunzionamenti e incidenti (*slopping*);

La risoluzione di tali criticità è assolutamente necessaria e urgente. Sono notevoli i ritardi anche nelle bonifiche che rappresentano ulteriore fonte primaria di inquinamento.

riportare le parole dell'ex presidente di Assindustria di Taranto, Antonio Caramia, un imprenditore, un industriale, il quale questo decreto ILVA se ne infischia di Taranto e dei tarantini: elargisce immunità ai nuovi acquirenti, senza offrire garanzie reali in tema di risanamento ambientale, mantenimento dei livelli occupazionali, piani industriali. La follia è arrivata a tal punto che, per pagare il fiume di soldi che lo Stato sta elargendo all'ILVA, potrebbe rendersi necessaria una stangata sulla bolletta elettrica. Questo è un elemento di grande rischio. Tutto questo ci convince ancora di più di una cosa: l'ILVA va chiusa. Va chiuso un ciclo industriale che produce malattie e morte (non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma gli industriali); va chiuso un modello che non dà più ricchezza e sviluppo al nostro territorio; va chiusa una realtà che non offre garanzie e stabilità occupazionali; va chiusa una fabbrica che produce debiti e inquinamento; va chiusa un'industria tenuta in vita artificialmente da undici decreti-legge. Il futuro di Taranto non può essere segnato dai *wind day*, dai giorni di forte vento, in cui il massimo che si può dire agli abitanti del rione Tamburi è: «Tappatevi in casa». Il prossimo passo quale sarà? Raccomandazioni sanitarie che consigliano di non respirare? È davvero troppo, siamo al colmo. La strada da percorrere è una soltanto: soltanto: abbandonare un risanamento impossibile per intraprendere nuove occasioni di sviluppo che puntino ad un sistema industriale innovativo e diffuso, alla valorizzazione della filiera agroalimentare e turistica, all'implementazione dei trasporti e della logistica.

dal dicembre del 2012 a oggi. Un insieme di norme che poco o nulla hanno risolto. Quest'ultimo decreto-legge reca disposizioni per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, ma i tempi per la cessione rischiano di diventare lunghi, anche perché le offerte presentate dalle due cordate che si affronteranno nella gara per l'acquisizione dello stabilimento di Taranto verranno sottoposte ad un gruppo di esperti, nominati dal Ministero dell'ambiente, i quali dovranno valutare la coerenza delle offerte con il piano ambientale. Non solo, quindi, il Governo ha ritenuto necessario affidare la gestione dell'ILVA a tre commissari straordinari, ma adesso ritiene opportuno attendere la validazione della commissione di esperti di esperti sulle offerte presentate. Ma non era sufficiente confidare sull'esperienza e sulla professionalità dei commissari straordinari, dal momento che conoscono la situazione in cui versa l'ILVA? No, per il Governo la soluzione migliore è quella di passare il testimone da un gruppo di esperti all'altro, con l'inevitabile conseguenza di rinviare a chissà quando la rinascita di un polo siderurgico di importanza strategica e di non risolvere i problemi connessi alla bonifica ambientale e alla salute dei cittadini. l'undicesimo decreto-legge che non aiuta a fare passi avanti; rappresenta, in buona sostanza, la proroga di una situazione di emergenza che ritengo non sia più ammissibile. Inoltre, si ravvisano nel contenuto di questo decreto-legge ulteriori e gravi profili critici e pochissime note positive. Con riguardo all'unico aspetto positivo che si intravede nel provvedimento, è da me condiviso l'emendamento approvato alla Camera che va a favore delle imprese dell'indotto, con il quale si è data priorità al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Non è, infatti, da sottovalutare che la questione non è circoscritta esclusivamente all'ILVA, ma attorno a questa si muovono centinaia di altre aziende, che basano la propria sopravvivenza e continuità economica esclusivamente sui rapporti commerciali e di fornitura con l'ILVA. Quanto alle criticità più rilevanti, è contrario a ogni logica giuridica e ai principi di un ordinamento che si basa sullo Stato di diritto, l'aver previsto uno scudo giudiziario che protegge gli acquirenti, affittuari e loro delegati in merito alle responsabilità connesse all'attuazione del piano ambientale dell'ILVA. Si tratta di un'estensione di uno strumento già in vigore per i commissari straordinari dell'ILVA e i loro delegati. La norma, contenuta in questo decreto-legge, prevede un'immunità

che si applica sino al giugno 2017 o, al massimo, fino al dicembre 2018, se vi è una proroga del piano ambientale. Ritengo che questa disposizione, che esclude dal regime di responsabilità i commissari, gli acquirenti e gli affittuari e i loro delegati, rappresenti un'anomalia giuridica di una gravità assoluta. È davvero singolare, nondimeno pericoloso, che, mediante un decreto-legge di diretta emanazione dell'Esecutivo, si pongano dei limiti all'azione giudiziaria e amministrativa con riferimento all'eventuale ipotesi di reato

per gestire la fase transitoria prima della cessione. Era stabilito, altresì, che l'acquirente avrebbe restituito il prestito, maggiorato degli interessi. in esame si paventa il rischio che queste somme finiranno per essere pagate, nella bolletta elettrica, dai cittadini italiani, i quali di colpo diventano finanziatori inconsapevoli. Tutto si sostanzia nel coinvolgimento della Cassa dei servizi energetici ambientali, che dovrà coprire gli oneri derivanti dai 300 milioni di euro versati a favore dell'amministrazione straordinaria nel 2016. La somma, per non incorrere nelle procedure di infrazione previste dalla legislazione europea in materia di aiuti di Stato, dovrà essere restituita entro il 2018, con il rischio evidente che verrà recuperata attraverso aumenti della bolletta elettrica. Un semplice ordine del giorno, approvato dalla Camera dei deputati, che impegna impegna il Governo, in caso di mancanza di cassa, a individuare le risorse necessarie per evitare eventuali aumenti nella bolletta degli italiani, non ci lascia certo tranquilli. È un dato di fatto che questo Governo ha preso di mira la bolletta elettrica per far pagare ai consumatori italiani imposte occulte. Ne è un esempio anche la decisione del Governo di imporre il pagamento del canone RAI, inserendolo coattivamente nella bolletta elettrica. Forza Italia, anche in quella occasione, ha espresso posizioni fortemente contrarie alle scelte del Governo, che non mancano di vessare noi cittadini con imposizioni fiscali sempre più elevate. In conclusione ritengo che sia del tutto inutile procedere ripetutamente con decreti-legge, su cui molto spesso, come in questo caso, viene apposta la questione di fiducia da parte del Governo. Non solo siamo di fronte al bieco atteggiamento dell'Esecutivo di neutralizzare ed esautorare le funzioni proprie del Parlamento, ma ancor di più non è possibile sostenerlo, dal momento che lascia immutata la situazione critica dell'ILVA di Taranto e non dà alcuna soluzione alle due priorità imprescindibili, ovvero il rilancio economico del polo siderurgico tra i più importanti d'Europa e la necessaria e improcrastinabile bonifica ambientale.

*vis* polemica si dimenticasse che da una parte c'è chi ha creato il problema e, dall'altra, chi oggi sta cercando di risolverlo. Mi colpisce anche la sottovalutazione della difficoltà di un'impresa come quella che si è proposta questo Parlamento e lo stesso Governo; è un'impresa veramente molto difficile. Per realizzare questa impresa credo sia giusto che il Governo e il Parlamento mettano in campo ogni strumento possibile per fare in fretta, per fare bene, per ottenere l'obiettivo che ci siamo dati fin dall'inizio: tenere in vita l'ILVA mettendo in campo tutti i mezzi per garantire salute e lavoro e mettendo al primo posto il risanamento ambientale e le bonifiche. Non è un caso che

un altro elemento: abbiamo dato tempo per valutare, insieme alle aziende che vogliono acquistare, le modalità e i percorsi per realizzare quelle prescrizioni, proprio per arrivare al risanamento ambientale. si è parlato di immobilismo. Ho sentito interventi che praticamente raccontavano che abbiamo cominciato oggi a occuparci di ILVA. Voglio ricordare che, grazie ai decreti-legge precedenti, sono già stati conclusi 112 degli interventi previsti previsti dall'autorizzazione integrata ambientale e altri 58 sono in corso, per cui si sta lavorando; non è vero che i decreti precedenti, proprio sul fronte del risanamento ambientale, non abbiano prodotto nulla.

Ci sono 11.000 lavoratori, 15.000 se contiamo l'indotto. C'è una questione che riguarda la politica industriale di questo Paese. questo Governo si è impegnato a salvaguardare un pezzo fondamentale dell'industria di questo Paese, quello siderurgico; lo sta facendo adesso su ILVA e l'ha fatto su Terni. Credo che lo Stato

L'altro aspetto, che vorrei non sfuggisse in questa discussione, è che il Governo di questo Paese su Taranto si è posto un altro obiettivo: rilanciare complessivamente la città. Dopodomani si inaugurerà il secondo piano del Museo archeologico di Taranto, uno dei poli museali più importanti del nostro Paese; è un investimento di questo Governo. Vorrei anche ricordare, ancora sul fronte occupazionale, che in questi giorni si sta discutendo del futuro di 520 lavoratori del porto di Taranto, dei

In questa discussione non ho sentito alternative; ho sentito accuse di retorica, ho sentito solidarietà al gruppo Riva. Ci dicano cosa vogliono fare e cosa avrebbe dovuto fare il Governo quelli che oggi ci dicono che le cose non

che cosa ne sarà di quei lavoratori, cosa ne sarà di quell'indotto. Ho sentito interventi appassionati. Ho sentito